o solare a concentrazione, è una tecnologia finalizzata allo sfruttamento dell'energia solare per generare energia elettrica. Attualmente, la pratica più diffusa è quella che utilizza dei collettori parabolici lineari. Da circa 20 anni sono in esercizio nove grandi impianti tipo in California e nel 2007 l'evoluzione delle procedure ha fatto sì che entrasse in servizio la prima centrale americana di nuova generazione. In Europa è stata la Spagna nel 2004 ad avviare un vigoroso programma industriale finalizzato alla realizzazione di una trentina di centrali di potenza complessiva di circa 1.300 megawatt. Nel 2007 il gruppo italiano Gengroup, specializzato per la produzione di energia da fonti rinnovabili, è stato incaricato della realizzazione in Libia della prima fase della costruzione di una centrale a ciclo solare termodinamico. Il sistema adottato è quello della struttura modulare con collettori parabolici lineari collegati in serie. Ogni collettore, costituito da un riflettore di forma parabolica, è in grado di concentrare i raggi solari cosicché il calore assorbito viene trasformato in vapore cui temperatura varia dai 390 ai 500 gradi centigradi. Le tecnologie più avanzate, che sono frutto

la condizione perché si sviluppi energia è la presenza di insolazione. Il sistema studiato in Italia dal gruppo riferentesi a Carlo Rubbia ha infatti introdotto una variante per cui, con l'applicazione di specifici sali, è possibile mantenere la temperatura

Un altro elemento positivo che si è manifestato nel corso di questi ultimi anni è l'abbattimento dei costi,

È ovvio che le potenzialità del solare a concentrazione termodinamica sono destinate ad aumentare se l'energia prodotta in Paesi a forte insolazione come l'Italia potesse essere esportata a regioni con una maggiore domanda e minore insolazione.

l'ENEA venne commissariata ed il professor Carlo Rubbia rinunziò a lavorare in Italia essendo stato con decreto governativo messo da parte il suo genio.

i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici;

Governo: ad adottare ogni iniziativa volta a promuovere la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici ad adottare ogni iniziativa finalizzata alla promozione delle energie rinnovabili, a porre in essere ogni atto di sua competenza volto a dare piena attuazione a quanto già previsto dalla legge finanziaria per il 2008 in materia di incremento dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, ad adottare ogni iniziativa volta a promuovere la formalizzazione di accordi di programma tesi a sostenere lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti e apparecchi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, dando effettivo seguito alle intese già

la recente approvazione del disegno di legge governativo recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha, a conclusione di un ampio dibattito parlamentare, definito il piano energetico nazionale prevedendo un programma di riassetto del *mix* delle fonti di produzione di energia necessario a sostenere l'elevato livello di domanda interna *pro capite*, tipico di un Paese sviluppato quale è il nostro, è il nostro, e le dinamiche di aumento della domanda che, superata presto come tutti ci auguriamo la crisi economica in atto, accompagnerà una nuova fase di sviluppo. La previsione normativa affronta tali prospettive tenendo presenti due obiettivi strategici essenziali: il primo è quello della riduzione della percentuale, attualmente attestata a circa l'88,4 per cento, di dipendenza da fonti di produzione energetica tradizionali o comunque non nazionali; il secondo è quello del rispetto degli accordi internazionali in materia di riduzione delle emissioni di CO2. Su questo secondo punto, tuttavia, il Governo ha già preso atto e in più sedi riferito della pratica impossibilità al mantenimento degli impegni imprudentemente assunti ha ottenuto in sede comunitaria alcune modifiche per settori della nostra industria, nonché una possibilità di revisione delle intese nel loro complesso, da discutersi dopo Copenaghen, nel marzo 2010, alla luce della direttiva di intenti scaturita dal dibattito al recente G8 in tema di cambiamenti climatici, che nel concreto ha preso atto della necessità di delineare in materia nuovi obiettivi e singoli piani d'intesa affrontabili da un indispensabile più ampio contesto di Nazioni. Ma su tale fondamentale materia, sulla ardita strumentalità e sfrontatezza di alcune previsioni, dovremo più ampiamente tornare a discutere a tempo debito. Governo e Parlamento hanno quindi stimato come corretto ed utile per il nostro Paese un equilibrio nella individuazione delle fonti energetiche, che preveda a regime l'utilizzo di quelle tradizionali non rinnovabili e di origine fossile (petrolio, gas, carbone) per non più di un 50 per cento del fabbisogno, del nucleare da nuove centrali di terza generazione per un ulteriore 25 per cento e di fonti energetiche rinnovabili per il rimanente 25 per cento. Il mantenimento della produzione di energia da fonti tradizionali non rinnovabili comporta comunque ed in ogni caso l'esigenza di una poderosa azione di rivisitazione e riconversione degli impianti più datati, per eliminarne l'effetto inquinante e quello ambientale devastante, a tutela della qualità della vita nei territori che li ospitano. li ospitano. Inoltre, per le nuove centrali nucleari, cercando di trarre in positivo il ritardo - con i suoi conseguenti costi - accumulato dal nostro Paese in materia, sarà utilizzata la più moderna tecnologia, in grado di assicurare la massima sicurezza ed il minimo impatto ambientale.

utilmente da scoprire), quanto sulle migliori tecnologie per un loro utilizzo in termini di efficacia, quindi per un migliore rapporto tra costi e benefici e - potrebbe apparire paradossale - in termini di impatto ambientale, caso variabile a seconda della fragilità del contesto paesaggistico e delle realtà geopolitiche e strutturali dei singoli territori. Nella nostra Italia, in particolare, dove l'incremento urbanistico ha già occupato spazi ampi e qualitativamente pregiati e e dove, soprattutto, le zone di interesse culturale, storico, paesaggistico sono così diffusamente presenti, sì da configurare quasi un unico pregiato contesto, patrimonio dell'intera collettività nazionale, ci si interroga maggiormente sull'opportunità di alcuni insediamenti a forte impatto. Le stesse intelligenze che anni or sono, nell'esigenza di contrastare i danni per inquinamento causati dagli impianti di produzione di energia tradizionali - i quali hanno compromesso, oltre alla salute di molti cittadini, importanti fasce costiere e zone di interesse ambientale del nostro Paese

all'interno della sempre più vasta gamma delle stesse rinnovabili, ma anche sul confronto con le nuove tecnologie delle non rinnovabili. Certamente, i progressi della ricerca scientifica, che assicurano - come dicevo - nuovi livelli di qualità per sicurezza ed efficienza, e la caduta, si spera, di residui pregiudizi ideologici consentiranno una possibilità di raffronto sereno ed oggettivo tra le tante opzioni energetiche, che alcuni anni addietro appariva impossibile. Premetto che il nostro Paese non è arretrato, come alcuni vorrebbero far credere, nell'utilizzo delle fonti naturali rinnovabili per la produzione di energia: è infatti il Paese, signor Presidente, che impiega il maggior quantitativo di incentivi per tali ed è, sotto non pochi profili, punta di eccellenza in tale campo. Anche in questo settore, allora, si impongono nuove scelte in ordine alle tecnologie da adottare, da incentivare e sulle quali concentrare ricerca e risorse. Occorre, in buona sostanza, che si elabori un piano complessivo e completo

costi, impatto sul paesaggio, continuità di erogazione, contenimento della dispersione in fase di trasmissione, capacità di incidere sul recupero di efficienza energetica dei settori che ancora nel nostro Paese costituiscono la maggiore causa di spreco (cioè l'edilizia e i trasporti). fattori che, non asetticamente o singolarmente pesati, debbono coesistere in un'unica complessiva valutazione - come dicevo - serena e oggettiva e possibilmente esente dall'influenza di pressioni industriali o finanziarie e anche scientifiche di parte, esorbitanti rispetto al vero interesse collettivo. Sottrarre a livello mondiale le decisioni in materia di energia alle pressioni industriali e finanziarie è certamente pura utopia (così come in molte altre materie), ma provarci, ognuno di noi per le proprie energie e competenza, credo sia dovere di tutti. Abbiamo cercato di affrontare con questi profili di realismo e oggettività anche il tema posto all'attenzione del Senato nella discussione di queste mozioni. della nostra mozione si intendono introdurre più ampie considerazioni che, come dicevo, dovremo in prosieguo di tempo più diffusamente sviluppare. Nella premessa si evidenziano invece alcune perplessità che, alla luce di quanto sino ad oggi accaduto, inducono a considerare con prudenza una massiccia diffusione di impianti a solare termodinamico nell'ambito del nostro territorio nazionale, ma non certo a non considerare positivamente l'utilizzo dell'energia solare, come alcuno ha strumentalmente voluto fraintendere. Infatti, i riscontri tecnici e maturati da esperienze in altri Paesi, per i cui dettagli rinvio al testo, portano a dire che un impianto di produzione termodinamica può essere installato solamente occupando grandi superfici, obbligate ad ampliarsi per ospitare le strutture di servizio e di stoccaggio e, quindi, richiede un attento esame di compatibilità paesaggistica e anche un consumo di risorse idriche non indifferente. Esso, tanto di installazione quanto di gestione, attualmente molto superiori a quelli di altre fonti energetiche, sia tradizionali che rinnovabili. E infatti, i Paesi che ne hanno attivato grandi impianti - si è citato l'esempio della Spagna sono costretti a un elevato e continuo esborso per le necessarie compensazioni sul mercato interno tra il costo dell'energia ordinaria e il costo dell'energia prodotta con quei sistemi, mentre altre Nazioni hanno addirittura dismesso quegli impianti. Per questo, alcune fasi del processo integrato di conversione e accumulo non registrano ancora significative attenzioni dal mondo della ricerca. Le disponibilità comunque stanziate dal precedente Governo con il decreto ministeriale dell'11 aprile 2008 non registrano richieste di utilizzo. Infatti, su 40 milioni vi sono solo tre progetti di preavviso, e non di richiesta di utilizzo, per un totale di 15 milioni, e nessuno di quei progetti ha ancora visto la sua definizione, o quanto meno la sua messa all'attenzione. Ciò lascia pensare ad uno scarso interesse dei possibili utilizzatori utilizzatori o, ancora di più, ad una cattiva elaborazione di quel decreto che avrebbe posticipato all'entrata in vigore degli impianti l'erogazione dei contributi,

la pur lodevole iniziativa degli stessi imprenditori). Quindi, comunque, quel decreto va sicuramente rivisto, quanto meno nelle sue modalità di utilizzazione dei fondi. I coefficienti di rendimento energetico non sono superiori a quelli di analoghe superfici che utilizzano altre tecnologie e per le quali la ricerca sta costantemente sviluppando processi di incremento e di redditività. Tutte queste criticità rendono ad oggi difficilmente compatibili (ma non impossibili), per caratteristiche di sostenibilità ambientale e di economicità, attivazioni di tali impianti sul territorio nazionale. Esse, per altro, non escludono certamente il fatto che possano essere compatibili con iniziative di grandissime dimensioni, da promuovere in territori diversi da quello europeo. Non è quindi da escludere che in zone del globo possano immaginarsi grandissimi impianti attivati con questa tecnologia, sfuggendo comunque - e questo sia chiaro - a facili suggestioni, come quella che essi possano assolvere alla domanda energetica del pianeta, ed assicurandosi che un ferreo patto internazionale di finanziamento e gestione degli impianti possa indurre a superare preoccupazioni strategiche legate alla localizzazione del sito di produzione. Diversamente, verrebbe meno anche l'effetto strategico della rivisitazione della politica energetica del nostro Paese. Concludendo, intendiamo sostenere la politica energetica recentemente definita dal Governo e dal Parlamento, che deve comunque, in sinergia con il settore privato, fortemente alimentare la ricerca scientifica e gli studi, valorizzando le intelligenze nazionali che nel tempo sono state sempre all'avanguardia nel mondo, e contribuire, con esse, sostanzialmente al dibattito internazionale sull'ambiente in tutte le sue sfaccettature,

il noto chiuso *club* dell'ambientalismo catastrofista che continua a sollecitare, sul fronte di una velleitaria lotta al cambiamento climatico, l'utilizzo di ingenti risorse pubbliche e quindi dei consumatori. Riteniamo che tali risorse ben più utilmente potrebbero essere destinate ad interventi di conservazione dell'ambiente, di riqualificazione del territorio (dalle risorse idriche ai dissesti idrogeologici), dell'edilizia e delle tecnologie nel settore dei trasporti, con particolare riferimento alla mobilità interna, nonché al sostegno della ricerca avanzata nella scoperta di nuove fonti pulite di energia, dalle quali potrebbero derivare grandi vantaggi. Riteniamo, come ho detto, indifferibile che il nostro Paese adotti un piano di promozione e utilizzo delle energie rinnovabili compatibile con le premesse di cui abbiamo sommariamente riferito in questa direzione si stanno già svolgendo i lavori della 13a Commissione, che ho l'onore di presiedere, nell'ambito di un'indagine conoscitiva sulle energie rinnovabili, che non mancherà di approfondire una oggettiva valutazione anche sulla tecnologia del termodinamico e sulle sue possibilità di di applicazione. Un dibattito che oggi è più che mai aperto e sul quale rivendichiamo, assieme alle Commissioni 7a e 10a, di avere coraggiosamente contribuito a sollecitare una nuova e più ampia riflessione. Molti di coloro che anni fa non avrebbero mai pensato di dover alimentare dubbi su alcuni dogmi del più ideologizzato ambientalismo sono oggi entrati in una fase di liberale ripensamento e di dialogo; hanno fatto, come si suol dire, macchina indietro, ad esempio sul nucleare. Siamo in attesa che anche le strutture governative siano in grado di superare l'imperante e comodo conformismo e mostrino la capacità di scendere sul terreno del confronto per un dibattito aperto, realistico commisurato ai più recenti progressi della ricerca scientifica e tecnologica, capace di interpretare le vere esigenze ambientali dei singoli territori e di dedicare attenzione alle loro specifiche necessità.

dell'umanità e in questa direzione è andato anche il recente vertice del G8. In tale sede, hanno assunto particolare rilievo i temi ambientali, sia a seguito del nuovo approccio americano alla lotta ai cambiamenti climatici, sia in conseguenza dell'approssimarsi di importanti scadenze scadenze politiche internazionali, quali il vertice di Copenaghen nel dicembre 2009 e la scadenza del Protocollo di Kyoto del 2012. Le conclusioni del vertice hanno messo in evidenza la consapevolezza che quello della lotta ai cambiamenti climatici è un tema globale e trasversale, che richiede risposte coordinate e, in maniera indissolubile, il coinvolgimento di tutti i Paesi, in primo luogo di quelli che sono i maggiori responsabili delle emissioni inquinanti. Le iniziative assunte negli ultimi mesi da parte del Governo degli Stati Uniti hanno messo in atto un netto cambiamento di rotta, confermando il carattere prioritario dei temi ambientali, anche durante la crisi economica, soprattutto a favore delle fonti rinnovabili di energia e di riduzione delle emissioni. Questa posizione è coerente con la strategia europea per un aumento dell'efficienza e della sicurezza energetica nel nostro continente, tenendo conto contestualmente della necessità della diminuzione delle emissioni che inquinano, e promuove l'incentivazione degli investimenti e delle azioni mirate all'incremento del contributo di energia da fonti rinnovabili rinnovabili e anche al miglioramento dell'efficienza energetica. L'Europa in questo contesto ha svolto un ruolo propulsivo sulla materia e le va riconosciuto il merito di aver affrontato, prima tra tutti, con l'accordo sul pacchetto clima/energia, clima/energia, la questione in termini concreti per trovare soluzioni equilibrate e sostenibili. Il cosiddetto Accordo europeo del «20-20-20» sul pacchetto clima-energia ha costituito un modello di riferimento a livello internazionale e un passaggio decisivo per indurre anche gli altri Paesi ad intraprendere la strada di un maggiore impegno nella lotta ai cambiamenti climatici ed, inoltre, ha fornito un contributo pratico alla strategia per l'abbattimento delle emissioni inquinanti e per il risparmio energetico senza pregiudicare le prospettive di crescita del sistema produttivo del continente. La maggiore sensibilità manifestata dall'Europa per il tema trae origine anche dalla condizione di precarietà che caratterizza il nostro continente, per quanto concerne gli approvvigionamenti energetici, per la minore disponibilità di fonti di energia e per la maggiore dipendenza da fornitori terzi. In questo quadro, l'obiettivo dell'incremento della produzione di energia pulita ma anche quello del risparmio e della maggiore efficienza nei consumi di energia assumono un rilievo veramente importante e particolare. Sono infatti noti gli sforzi che devono fare gli Stati membri ed in particolare l'Italia per ottemperare al cosiddetto Accordo del 20-20-20, specialmente nell'attuale momento di crisi economica e finanziaria abbattutasi sul sistema globale, che richiede un'assunzione di responsabilità circa le politiche da mettere in atto per difendere e rilanciare l'economia globale. La compatibilità ambientale e il risparmio energetico stanno diventando elementi strutturali delle politiche economiche, dei processi produttivi, delle politiche abitative e della mobilità. Si offre l'opportunità per avviare una fase di trasformazioni radicali nelle tecniche di produzione, attraverso la riconversione di alcuni comparti e lo sviluppo di nuovi settori produttivi. Investire in efficienza energetica consente di alleggerire, in tempi relativamente brevi, i costi energetici a carico delle famiglie e delle imprese. Promuovere un maggiore sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili può avere - come come ha già avuto in altri Paesi - conseguenze positive sul piano dell'occupazione, dell'innovazione tecnologica e dell'affermazione di nuovi settori industriali, al tempo stesso ad alto contenuto di tecnologia e ad elevata intensità di lavoro. Il nostro Paese ha recepito la direttiva 2001/77/CE, relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, che costituisce la base legislativa per promuovere la produzione di elettricità attraverso il contributo delle fonti energetiche rinnovabili, tra le quali anche il solare termodinamico.

ai fini dell'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante impianti solari termodinamici, anche ibridi, tale decreto ha previsto, in favore delle persone fisiche e giuridiche responsabili degli impianti, tariffe incentivanti per un periodo di 25 anni per l'energia elettrica prodotta; negli ultimi anni la tecnologia del solare termodinamico o solare a condensazione ha raggiunto rilevanti progressi e innovazioni che permettono di accumulare il calore prodotto e renderlo disponibile quando richiesto, eliminando la variabilità di rendimento che ha sempre caratterizzato questi impianti limitandone le potenzialità di sviluppo; l'aumento dell'efficienza energetica e la progressiva riduzione dei costi iniziano a rendere questa tecnologia competitiva rispetto a quella dei combustibili fossili; secondo il rapporto preliminare sullo stato attuale del solare termico nazionale, redatto dalla Commissione nazionale per l'energia solare, le prospettive di mercato prevedono una riduzione del costo livellato degli impianti che sfruttano il solare termodinamico, dagli attuali 16 USc/KWh a circa 6 USc/KWh, entro il 2025, raggiungendo a tale data il costo previsto per gli impianti a combustibile fossile; altre fonti prevedono costi addirittura inferiori, fino a 3,5 USc/KWh; si tratta di una tecnologia che interessa soprattutto i Paesi a forte insolazione, come il nostro, tuttavia, gli impianti esistenti nel mondo sono tutti costruiti in zone desertiche, in considerazione dell'ampio spazio necessario per lo sviluppo dei collettori parabolici lineari, collegati in serie, che rappresentano la grande maggioranza di tali impianti; lo sviluppo del solare termodinamico nel nostro Paese deve tenere conto delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi di intervento, in considerazione dell'importanza che riveste la qualità del paesaggio per l'attrattività turistica e per l'economia nazionale; la recente approvazione dal Parlamento del disegno di legge del Governo recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia crea le condizioni per l'avvio di programmi coerenti con quelli comunitari in materia di energia nucleare ed incentiva la produzione di energia da fonti rinnovabili permettendo al Paese di di recuperare quel *gap* energetico accumulato negli anni nei confronti dei Paesi più all'avanguardia, impegna il Governo: a promuovere lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili per la produzione di energia elettrica, consolidando meccanismi di incentivazione coerenti con le più avanzate esperienze europee; europee; a sostenere, parallelamente con lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, tutte le azioni occorrenti per l'avviamento di programmi coerenti con quelli comunitari in materia di energia nucleare,

ambientale; ad adottare nell'ambito della promozione delle energie rinnovabili ogni iniziativa utile allo sviluppo della ricerca per il perfezionamento ed il miglioramento dell'efficienza energetica nel settore dell'energia solare fotovoltaica, di quella eolica,

principalmente nel settore dell'edilizia ed in quello dei trasporti che tuttora costituiscono i settori a maggiore dispersione energetica del Paese; a destinare ai suddetti obiettivi tutte le possibili risorse, ivi comprese quelle dei fondi non attivati per l'incentivazione di energie non ritenute proficue; non ritenute proficue; a privilegiare lo strumento degli accordi di programma sui progetti in ricerca e tecnologia indirizzati allo sviluppo di attività per la produzione di impianti e apparecchi per le fonti rinnovabili utili a sostenere l'efficienza del mondo produttivo e l'economicità dei consumi dei privati cittadini.

la mozione del Gruppo del PD vuole richiamare l'attenzione su un'importante fonte di energia alternativa con moltissime possibilità di sviluppo. In generale, lo sviluppo dell'intero settore delle energie cosiddette alternative rinnovabili ci vede fortemente interessati e la promozione della ricerca in questo campo è per noi fondamentale. In particolare, vogliamo oggi sottolineare i significativi progressi che abbiamo avuto, proprio grazie a studi e tecnologie italiane, nel campo del solare a concentrazione o solare termodinamico, che produce calore ed elettricità usando centinaia di specchi per concentrare i raggi del sole ad altissime temperature. È ovvio che un Paese come il nostro sia interessato, ed è altrettanto facile comprendere i benefici che l'Italia può trarre da questo tipo di energia e da moltissime applicazioni e tecnologie in rapido sviluppo, destinate a renderci meno legati ad altri Paesi per l'approvvigionamento energetico e ad avere progressivamente un buon rapporto tra produzione e costo. Tale tipologia energetica è in fase di espansione. Alla fine del 2008 le centrali solari a concentrazione hanno raggiunto una potenza di 436 megawatt in tutto il mondo ed entro il 2011 la potenza, grazie ai progetti in corso, soprattutto in Spagna, sarà quasi triplicata; nel 2017 gli Stati Uniti e ancora la Spagna avranno ulteriormente esteso e moltiplicato la produzione di energia da solare a concentrazione. Nel 2030, da alcune parti si stima che il solare a concentrazione fornirà il 7 per cento circa dell'elettricità mondiale,

Sempre secondo questo scenario più moderato, il settore svilupperà nel 2020 oltre 200.000 posti di lavoro nei Paesi più esposti a radiazione solare, fino a raggiungere 1.100.000 posti nel 2050. Avremmo invece il raddoppio dei posti se si verificasse lo scenario di sviluppo più avanzato. Gli investimenti per conseguire tali risultati sarebbero assolutamente ragguardevoli: 36 miliardi di euro nel 2020 e 92,5 miliardi di euro nel 2050 sullo scenario moderato; 40 miliardi di euro nel 2020 e 174,5 miliardi di euro nel 2050 secondo lo scenario di sviluppo avanzato. Il risparmio di CO2 sarebbe almeno di 2,2 miliardi di tonnellate annue, pari a circa quattro volte le emissioni attuali dell'Italia. Il costo di produzione, come si diceva, va diminuendo e diverrà competitivo, secondo molti operatori, rispetto a quello delle centrali a gas. In Italia abbiamo importanti progetti che già si sono concretizzati e che stanno generando nuove possibilità operative. È il caso del progetto Archimede di Priolo Gargallo (Siracusa), che vede all'opera la presenza e l'intelligenza del professor Rubbia e sta raggiungendo costi accettabili per la produzione energetica, destinati a scendere ulteriormente. Peraltro, già negli Stati Uniti i costi di produzione energetica in impianti di nuova generazione sono diminuiti negli ultimi 10-15 anni, e presto scenderanno sotto i cinque centesimi di dollaro per chilowattora. Le possibilità di sviluppo e di applicazione sono molteplici, soprattutto se si considerano gli impianti a tecnologia ibrida, cioè quegli impianti che combinano tra loro diverse forme di energia che possono essere utilizzate contemporaneamente o sostitutivamente, favorendo il pieno e continuo approvvigionamento energetico. Tra le nuove possibilità di impianti combinati con sfruttamento contemporaneo di diverse forme di energie rinnovabili, cito l'esempio (se ne potrebbero fare altri) impianti modulari a tecnologia ibrida che sposano solare termodinamico e biomasse, con notevoli benefici. Ne ricordo alcuni: la possibilità di supportare l'evoluzione dei sistemi agro-energetici territoriali basati sulle coltivazioni di biomasse da "filiera corta" e da manutenzione boschi; delle emissioni di CO2; l'aumento della certezza dell'approvvigionamento energetico; l'incremento del livello di accettabilità sociale di cui gli impianti di produzione energetica in genere scarseggiano; l'aumento dell'efficienza energetica e dello sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili al minor costo possibile; ottenere un miglioramento delle condizioni ambientali a livello locale; il conseguimento, dopo un periodo di sperimentazione di speciali colture agroenergetiche, di un possibile disinquinamento di terreni agricoli inquinati. Questi erano solo alcuni esempi. Ancora, il solare a concentrazione è il fulcro di progetti di ricerca assolutamente rilevanti da parte di aziende leader del settore energetico: il Desertec è uno di questi e pone tecnologia e deserti al servizio della sicurezza energetica, idrica e climatica. Da ciò è scaturita l'idea della realizzazione nel deserto del Sahara di un impianto solare termico a concentrazione con una potenza di circa 100 gigawatt. Su Desertec la Germania ha orientato attenzione ed una massa consistente di investimenti. Sottolineo solo un elemento per dare l'idea della rilevanza di tali progetti: una superficie inferiore allo 0,3 per cento dei deserti nordafricani, ricoperta da specchi solari a concentrazione, sarebbe in grado di coprire i fabbisogni elettrici e di acqua potabile di una popolazione pari a quella Medio Oriente e del Nord Africa. Anche in questo caso, l'uso combinato di energie da fonti rinnovabili (ad esempio, eolico e solare a concentrazione) produrrebbe risultati eccezionali, senza impoverire il pianeta, all'insegna di quello sviluppo sostenibile che è ormai diventato necessità inderogabile per il mondo intero, consentendo una vita dignitosa a tanti popoli oggi esclusi dalla scena mondiale. Non è un'utopia! Servono capacità di guardare lontano, investimenti, progetti ambiziosi e lungimiranti, Governi che comprendano che la nuova economia e il futuro stesso dell'economia passano di qui. Avere la possibilità di produrre energia senza inquinare, da fonti rinnovabili, a prezzo contenuto, liberandoci da rapporti in politica estera talvolta equivoci, non è cosa da poco! Anche l'Italia è presente in questo scenario che abbiamo appena delineato. È italiana l'unica azienda al mondo che produce tubi ricevitori di vetro per sali fusi, elemento fondamentale dell'intero processo. Vi sono poi altre aziende italiane che portano avanti progetti simili basati però su tubi ricevitori a più basse temperature. La tecnologia in uso è stata sviluppata e brevettata nei laboratori ENEA di Portici. Molti sono i progetti avviati, grazie anche a un sistema di incentivazione introdotto dal Governo Prodi. ENEL a Siracusa sta realizzando l'impianto sperimentale del progetto Archimede; il programma Industria 2015 vede il finanziamento di due progetti, uno per lo studio di tubi ricevitori solari, l'altro per lo sviluppo della tecnologia solare termodinamica a concentrazione tramite specchi di tipo Fresnel. Si tratta di una tecnologia diversa da quella attualmente in uso. Ciò che è avvenuto in questi anni nel settore del solare fotovoltaico deve in qualche modo esserci di guida e segnare la nostra esperienza per anticipare mosse strategiche per il sistema Paese: è la tecnologia italiana che deve spingerci a queste riflessioni. Se guardiamo all'esempio precedente del solare fotovoltaico vediamo che la Germania, che per prima era partita nell'incentivare il fotovoltaico, oggi non è più solo leaderper numero di impianti installati, ma è anche leader nell'industria della componentistica fotovoltaica e le sue imprese utilizzano gli analoghi e successivi incentivi che gli altri Paesi europei hanno deliberato, spesso seguendone le tracce. Il risultato diretto è stato più occupazione interna e più esportazione di beni negli altri Paesi. C'è un precedente, dunque. Non vogliamo seguirlo? Anche in Italia oggi si sono sviluppate e rafforzate delle piccole realtà imprenditoriali lungo tutta la filiera, che hanno fatto del fotovoltaico la loro attività principale, ma la Germania ha usufruito in partenza di un notevole vantaggio. Questa volta il vantaggio potrebbe averlo l'Italia sul solare a concentrazione. Allora proprio questo deve essere l'obiettivo italiano per il settore del solare termodinamico: incentivare oggi per primi l'avvio della filiera per essere leader ed esportatori di tecnologia domani. Sempre guardando al *case history* precedente, quello del fotovoltaico, la seconda considerazione è la seguente: gli incentivi sono ben spesi! Infatti la logica dell'incentivo per avviare il mercato è risultata corretta, e oggi, a due anni dall'entrata in vigore del cosiddetto Nuovo Conto Energia voluto dall'allora Ministro dello sviluppo economico, Pierluigi Bersani, si sono installati in Italia ulteriori 390 MW, colmando in parte il *gap* con altri Paesi, ed i prezzi della componentistica si sono ridotti, per effetto della concorrenza e dello sviluppo del mercato, di quasi il 15 Sostenere dunque oggi il solare termodinamico con incentivi, ma anche facilitando la realizzazione di alcune centrali significative, vuol dire assicurarsi un primato tecnologico, e l'Italia può farcela; vuol dire avere per primi le riduzioni di costo della tecnologia, e quindi la riduzione di costi della produzione energetica; vuol dire, domani, far beneficiare la nostra industria degli incentivi che verranno promossi negli altri Stati. Un'ultima considerazione: a differenza di altre fonti rinnovabili, il solare termodinamico, opportunamente sviluppato anche in forme ibride, può realmente dare un contributo significativo sia in termini di potenza sia di energia prodotta per coprire i fabbisogni di elettricità del nostro Paese. Il grande interesse del sistema Paese risiede proprio nel fatto di essere ai vertici della conoscenza tecnologica in questo settore, esportata già per applicazioni in altri Stati, e sarebbe auspicabile che venissero realizzati più impianti italiani, oltre a quello di Siracusa. A questo punto, come non chiedere al Governo una politica più incisiva, che promuova con opportuni meccanismi di incentivazione lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili per la produzione di energia elettrica, unita ad impieghi non elettrici come la produzione di calore, la desalinizzazione dell'acqua del mare, la climatizzazione estiva? Come non chiedere, ancora, una politica volta a prendere seriamente in considerazione l'accordo comunitario con l'obiettivo cosiddetto del 20-20-20, che dia impulso all'intero settore del solare, dalla ricerca alla produzione, coinvolgendo tutto il sistema industriale e valorizzando i nostri centri di ricerca, le cui scoperte e le cui innovazioni tecnologiche sono tanto apprezzate all'estero? Una politica che incentivi i cittadini a scelte virtuose di risparmio energetico, coinvolgendo in particolare il settore dell'edilizia e quello dei trasporti, che costituiscono attualmente il maggior problema per lo spreco energetico e le sue nefaste conseguenze. Una politica infine, ma non da ultimo, che scelga di sostenere le imprese italiane, con un occhio di riguardo a quelle medie e piccole, che costituiscono l'ossatura del nostro sistema economico e che sono disposte a investire su produzione di energia da fonti rinnovabili o che contribuiscano all'incremento dell'efficienza energetica. Forse, con una politica così faremmo davvero un passo decisivo in campo ambientale verso un futuro dove la sostenibilità ambientale rappresenti un obiettivo raggiunto per tutti gli abitanti del pianeta - qui non si vince da soli e dove infauste previsioni di distruzione dell'ecosistema globale non trovino più alimento e non destino angoscia e paura quando si guardi al domani.

Onorevole Presidente, indubbiamente l'illustrazione delle

all'energia rinnovabile rappresentata dallo specifico settore del solare a ciclo termodinamico (è di questo che stiamo parlando), nella mozione illustrata dal senatore D'Alì si vuole impegnare il Governo esattamente nella direzione opposta, ossia, come si legge nel dispositivo, "ad adottare nell'ambito della promozione delle energie rinnovabili ogni iniziativa utile allo sviluppo della ricerca per il perfezionamento ed il miglioramento dell'efficienza energetica nel settore dell'energia solare fotovoltaica, di quella eolica, di quella proveniente dalle biomasse" e di quella connessa allo sfruttamento del mare. Non viene quindi citata l'energia rinnovabile del solare termodinamico. il Governo "a destinare ai suddetti obiettivi tutte le possibili risorse, ivi comprese quelle dei fondi non attivati per l'incentivazione di energie non ritenute proficue". Ossia si dice: anche i fondi che possono essere destinati destinati alla produzione di energia solare con ciclo termodinamico vanno invece destinati alle altre fonti rinnovabili. L'argomento in discussione in questa giornata non era quello delle energie rinnovabili, ma di una specifica energia rinnovabile,

il senatore D'Alì di destinare ad altre fonti rinnovabili i fondi esistenti.

«a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa volta a promuovere la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante cicli termodinamici, per i possibili sviluppi di tale tecnologia sia a livello nazionale che internazionale, provvedendo alla definizione di ulteriori ed opportune forme di incentivazione, nonché all'implementazione di quelle già definite».

la maggioranza propone una mozione che va in senso contrario rispetto a ciò che il Governo lo scorso 8 luglio ha ritenuto di condividere.

che nei locali del Parlamento italiano, a Palazzo San Macuto, nella Sala del Refettorio il 16 luglio scorso (una settimana fa) la Germania abbia presentato il progetto Desertec,

viene presentato nei locali offerti dal Parlamento italiano e noi restiamo a guardare,

è frutto del nostro genio, è il nostro progetto, è il progetto ENEA*,* è il progetto portato avanti dal professor Rubbia, che vedrà la sua realizzazione in altri Paesi. La Germania dunque diventa capofila di questo enorme progetto, che riguarderà la Libia, il Marocco e la Tunisia;

ha studiato il problema e, a proposito dei costi e con riferimento alla riduzione dei costi d'impianto in che, rispetto alla realizzazione in Sicilia dell'impianto Archimede da 5 megawatt, i costi di investimento già mostrano una netta tendenza alla riduzione, soprattutto per quanto riguarda i componenti tipici del campo solare, in virtù della maturazione dei processi di fabbricazione e dell'ottimizzazione dei progetti. Aggiunge, inoltre che le prospettive di applicazione nel medio-lungo termine in Italia dovrebbero riguardare la realizzazione di un impianto da 50 megawatt in ciascuna Regione del Sud, per un totale di circa 200 A livello internazionale le potenzialità sono molto più ampie. Le analisi internazionali indicano al 2020 una capacità installata complessiva di oltre 10.000 megawatt. La tecnologia italiana, dal punto di vista qualitativo, è già in posizione di vertice potendo vantare prestazioni altamente competitive. Sarà perciò necessario favorire un maggior sviluppo industriale in questo settore, stimolando la formazione di grossi raggruppamenti in grado di competere anche dal punto di vista della capacità produttiva. Questo lo dice il nostro ente di ricerca sulle energie rinnovabili

titubanza o addirittura proponiamo di disincentivare gli aiuti per il solare a ciclo termodinamico, destinando le risorse ad altre energie rinnovabili. Come non cogliere l'enorme occasione che all'Italia viene offerta, essendo Paese leader nelle conoscenze, nella progettazione e nella realizzazione della componentistica? Sono nostre le imprese che lavorano in Libia Libia e nostri i tecnici impiegati in Spagna e nel Nevada, così come sono componentistiche realizzate nelle industrie italiane quelle che vengono montate negli impianti del resto del mondo. E noi stiamo a guardare: è una sfida enorme alla quale siamo chiamati.

colleghi, nel contesto dell'obiettivo europeo di utilizzo del 20 per cento di fonti rinnovabili, rispetto al 1990, entro il 2020, l'Italia ha l'obiettivo nazionale del 17 per cento del consumo finale di energia da fonti rinnovabili, rinnovabili, pari a 28 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. Nel *position paper* italiano del settembre 2007, il potenziale teorico di rinnovabili stimato è di soli 24,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio. L'obiettivo europeo a cui siamo impegnati è dunque superiore persino alle stime teoriche e ottimistiche di sviluppo delle fonti rinnovabili definite dal Governo Prodi nel settembre 2007. In ogni caso, in quel documento, i 24,5 milioni di tonnellate equivalenti stimati erano suddivisi in 9 milioni di tonnellate, equivalenti a 104 terawattora di energia elettrica da rinnovabili, 9,3 milioni milioni di tonnellate di energia termica da biomassa, 4,2 da biocarburanti e 2,1 di energia termica da solare e geotermica. È opportuno evidenziare che una riduzione del consumo finale attraverso l'aumento dell'efficienza energetica superiore al *target* fissato, peraltro non in via perentoria, del 20 per cento, potrebbe consentire di ridurre l'obiettivo di produzione da rinnovabili al di sotto del potenziale stimato che noi - come si evidenziava prima - non saremmo comunque in grado di raggiungere. Peraltro, l'efficienza energetica negli usi finali è l'opzione più conveniente in termini di costi-benefici per la riduzione dei gas serra e, soprattutto, della dipendenza energetica del nostro Paese.

abbastanza diffusa. o ancora ad oltre 3000 centrali a biomassa da 2,5 MW, anch'essa una taglia che può considerarsi abbastanza diffusa. Per non parlare poi dei pannelli fotovoltaici, che richiederebbero per fornire questa quantità di energia

Oggi il costo di incentivazione delle rinnovabili, al netto delle fonti assimilabili, è di circa 1,6 miliardi di euro l'anno, una cifra che si prevede in crescita fino ad arrivare a 7 miliardi di euro nel 2020.

La politica energetica del Governo ha l'obiettivo di passare dalla situazione attuale, con oltre il 74 per cento di energia prodotta da fossili, l'11 per cento da fonti rinnovabili, e in gran parte dall'idroelettrico, e un restante 15 per cento da energia importata, principalmente dagli impianti elettronucleari francesi, ad uno scenario

di una serie di fattori o criteri tra i quali la convenienza economica, e quindi la minore necessità di incentivazione, l'indipendenza energetica, e quindi la disponibilità sul territorio nazionale della fonte, la cogenerazione di energia elettrica e termica, la compatibilità degli impianti con le caratteristiche paesaggistiche e geomorfologiche del nostro territorio, la presenza di *know how* e filiere produttive ed impiantistiche disponibili o sviluppabili all'interno del sistema industriale nazionale, la non competizione della fonte da sostenere con le produzioni alimentari ed il massimo sfruttamento degli scarti e dei rifiuti. Un elemento da valutare poi con grande attenzione è che il finanziamento delle politiche di incentivo delle rinnovabili non ricade sulla fiscalità generale bensì sui consumatori elettrici, con evidenti profili di iniquità contributiva per cittadini e aziende. Un ultimo aspetto da considerare nel fare le scelte di incentivazione è l'opportunità di sostenere lo sviluppo di competenze tecnologiche ed impiantistiche, così come nel nucleare anche nelle rinnovabili, fine di acquisire commesse sui mercati internazionali da parte dei nostri settori produttivi nazionali. La presenza di significative esperienze industriali nel settore dell'impiantistica, delle tecnologie dei fluidi, dei gas e del vapore, unita all'esigenza di riconvertire parte della capacità ingegneristica e produttiva di settori quali l'*automotive,* deve essere tenuta in debita considerazione. Per questi motivi le politiche di sostegno e di incentivazione della ricerca, del trasferimento tecnologico e dell'industrializzazione di sistemi innovativi di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili possono anche prendere in considerazione soluzioni non ottimali per il territorio nazionale, come l'eolico o il solare termodinamico, ma interessanti ed adatte a mercati in sviluppo come il Nordafrica verso i quali creare le condizioni ottimali per un'espansione commerciale e industriale del nostro sistema produttivo. Occorre evitare il pregiudizio negativo o positivo rispetto alle singole e diverse opzioni e considerare in ogni caso l'esigenza di mettere a punto un sistema di incentivi sufficientemente stabile, in grado di garantire i piani finanziari degli investimenti, ma al tempo stesso rapidamente adattabile alle evoluzioni tecnologiche e all'ottimizzazione dei costi industriali che naturalmente le dinamiche di mercato producono. Per queste ragioni riterrei molto utile valutare la possibilità di considerare le mozioni oggi in discussione un primo approccio dell'Aula del Senato ad un tema così complesso e strategico per il Paese, riservando il tempo necessario ad un ulteriore ed attento approfondimento tecnico ed economico del panorama delle opzioni tecnologiche presenti nel settore delle rinnovabili prima di formulare nuovamente indirizzi definitivi per il Governo. Peraltro, la Commissione ambiente sta completando un'indagine conoscitiva sulle energie rinnovabili e si appresta a predisporre un documento finale che potrebbe rappresentare un punto di vista più ampio sull'argomento oggi in discussione, in grado di tener conto del dibattito che si sviluppa in Aula e di un opportuno e approfondito confronto con la Commissione attività produttive, che ha certamente titolo e competenza per entrare nel merito di questo importante e delicato problema per lo sviluppo e per il futuro del nostro Paese, per le tecnologie, per l'economia e per l'ambiente.

economico*. Prima di esprimere il parere del Governo, vorrei svolgere alcune considerazioni, dal momento che il dibattito che si è sviluppato in quest'Aula - e ringrazio tutti i colleghi che lo hanno animato - riguarda un tema particolarmente rilevante. La discussione

Il Governo desidera sottolineare con forza l'impegno profuso in questi mesi, peraltro in linea con il lavoro già svolto dal Governo Berlusconi dal 2001 al 2006 Il rinnovato impegno su questo argomento è stato riproposto con l'approvazione, da parte del Parlamento, della cosiddetta legge sviluppo. Assieme alle fonti rinnovabili abbiamo costruito un sistema che siamo convinti potrà dare risultati anche sul piano dell'efficienza e del risparmio energetico. Per queste ragioni pensiamo che la linea del Governo sia perfettamente parallela

In particolare, riteniamo che per il solare termodinamico ci sia una serie di criticità, che il senatore D'Alì ha sottolineato, ma non pensiamo di privarci di questa opportunità, tenuto conto che l'implementazione di impianti a solare termodinamico nel nostro Paese oggi c'è un unico cantiere aperto, quello relativo - come è stato ricordato dal senatore Li Gotti - al progetto Archimede di Siracusa, promosso dall'ENEL.

Non abbiamo un pregiudizio ideologico nei confronti di alcuna fonte energetica. Pensiamo che il *mix* delle nostre fonti energetiche debba essere meno squilibrato nei confronti degli idrocarburi, e in particolare del gas, e che il contributo delle fonti rinnovabili sia decisivo.

del programma Industria 2015, in particolare quelli relativi alla innovazione tecnologica. Per tale ragione, pensiamo che questi strumenti debbano essere armonizzati con gli strumenti e gli incentivi anche per la realizzazione di nuovi progetti e con i finanziamenti europei, che in questo settore ci vedono protagonisti. Per quanto riguarda il solare termodinamico, vediamo una possibilità di implementazione, insieme ad altri Paesi (in particolare Francia e Germania), in tutta l'area del Mediterraneo. Si è fatto precedentemente riferimento a questi progetti,

perché evidentemente c'è ancora una necessità di approfondimento nella loro applicazione industriale. Non vi è quindi alcuna intenzione da parte nostra di ridurre o cancellare la ricerca e l'investimento in questo tipo di di tecnologie, ma siamo anche consapevoli, come del resto dice la mozione della maggioranza, che ci sono molte, molte criticità. Va anche tenuto conto di un altro aspetto: incontrando gli operatori delle industrie (che ovviamente debbono avere una certa dimensione per investire in questo tipo di tecnologie), ci viene sempre detto - credo a ragione - che anche gli impianti di solare termodinamico si reggono se associati a impianti termoelettrici tradizionali, tant'è vero che anche il progetto Archimede è basato su questo presupposto. C'è quindi la combinazione tra una